Domani, 7 novembre, l'Unione regionale delle Province siciliane, un organismo che aderisce all'Unione delle province italiane e che è prettamente istituzionale, ha organizzato una manifestazione a piazza Montecitorio, luogo idoneo e consueto di tante manifestazioni politiche, per richiedere l'applicazione - più volte sbandierata, ma mai avvenuta - di una norma della scorsa finanziaria che prevedeva il finanziamento

oggi ci informa che la manifestazione non può tenersi a piazza Montecitorio, ma deve essere spostata in altra sede. È un atto assolutamente inaccettabile! Non vorrei che a Roma il nuovo clima di sgomberi,

Cercherò nel tempo concessomi di esprimere una riflessione di merito sulla finanziaria utilizzando, in particolare, la rigorosa riflessione culturale e politica del Presidente della Commissione bilancio, il senatore Morando. Prima però vorrei fare una considerazione di ordine generale utilizzando una riflessione, a mio avviso, attenta, puntuale ed importante della senatrice Menapace, la quale, intervenendo nel dibattito, faceva riferimento... *(Brusìo).*

la quale faceva riferimento al governo della complessità e all'esigenza che abbiamo oggi di guardare complessivamente all'intreccio dei problemi. Ora, proprio Ora, proprio questo riferimento, che utilizzo un po' forzatamente e polemicamente, senatrice Menapace, mi consente di partire con un'affermazione. Questa finanziaria è un provvedimento coalizionale, non nel senso della capacità di esprimere la sintesi della complessità, ma come somma disorganica delle diversità e delle contraddittorietà. Lo conferma la dispersione e la frantumazione delle risorse di una finanziaria tutta chiusa nella dimensione del presente,

Il Mezzogiorno è una questione disattenzionata non soltanto attraverso questa finanziaria, è una questione di lungo periodo che riguarda trasversalmente le forze politiche e gli schieramenti.

È una finanziaria che rispetto al Sud riduce ancora di più il tema delle zone franche urbane e che non è capace di affrontare la grande questione della leva urbana come crescita per lo sviluppo del Mezzogiorno. È una finanziaria che non affronta alcuni nodi. Non basta, per questo faccio riferimento al suo intervento, ritenere che l'incentivo all'occupazione, cioè il *bonus* occupazionale correttamente diversificato nel caso di occupazione femminile, risolva il problema, soprattutto se si aggiunge che tale *bonus* occupazionale trova copertura finanziaria sui fondi del FAS e quindi, sostanzialmente, rappresenta una sorta

ad una manovra, a delle scelte, a dei provvedimenti - ad iniziare dal Protocollo sul *welfare* e sulla competitività - che guardano ai già garantiti, a soggetti che proteggono ulteriormente; basta fare riferimento, signor Presidente, ai dati contenuti nel libro di Tito Boeri «Contro i giovani.

cui, per ogni euro speso per chi ha meno di trent'anni, se ne spendono 3,5 per chi ha più di 65 anni, ci troviamo cioè in un Paese in cui bisognerebbe riequilibrare complessivamente la spesa. Invece il Governo,

perché correttamente la questione salariale andava inserita all'interno del Protocollo sul *welfare* e sulla competitività, non può essere un tema ed un elemento a venire.

proviene rispetto al 2008, di finalizzare le risorse recuperate per intervenire sul versante del lavoro dipendente, ma non c'è la concretezza delle scelte, di un impegno che - ripeto - a mio avviso, doveva trovare corretta collocazione all'interno del Protocollo sul *welfare*, perché è evidente che è in questo modo che si possono complessivamente affrontare le situazioni che abbiamo di fronte. Ci troviamo dinanzi ad una scelta che interviene esclusivamente in termini di risorse finanziarie sul tema dello scalone e solo a questo destina la straordinaria parte delle risorse complessivamente a supporto dell'articolo 62 della legge finanziaria per l'attuazione del Protocollo sul *welfare*. Il resto è poca cosa: rimodulazione dell'indennità di disoccupazione, interventi rispetto a due fondi da cento milioni di euro; restano tagliati sostanzialmente fuori i veri precari e non si affronta organicamente il tema delle nuove tutele, perché anche il *welfare* e il Protocollo sul *welfare* e la competitività stanno dentro la linea della tutela dei già garantiti e non della capacità d'affrontare un organico disegno di costruzione di nuove tutele. Basti pensare che tutto l'universo dei Co.co.pro. è sostanzialmente fuori dall'attenzione del Protocollo, tant'è che vi è il paradosso di lavoratori subordinati o a tempo determinato che hanno tutele e garanzie piene o ridotte e un intero universo di soggetti, quello dei veri precari, che non hanno alcuna garanzia, alcuna tutela, perché sono i soggetti assenti sul piano dell'attenzione del Governo di centro-sinistra. Mi rendo conto

Da tempo, sono convinto che la crisi della politica stia nel fatto che nessuno più si chieda: «Che cosa serve al mio Paese, che cosa serve alla mia Patria?». questa finanziaria non risponde alle esigenze di crescita e sviluppo del Paese; è dentro la crisi della politica e, per certi versi, la accentua: la crisi della politica, infatti, è incapacità di dare risposte, di compiere scelte coraggiose e di avere la forza di una visione. L'unica visione che emerge dalla finanziaria è quella di una coalizione frantumata, che non poteva che produrre

per la verità abbiamo visto anche un contributo importante dell'opposizione ed abbiamo raggiunto una importante soddisfazione, se è vero, com'è vero, che - a differenza dello scorso anno - siamo riusciti ad approvare un testo

dalla politica della pubblica amministrazione; la salvaguardia dell'incremento dei salari delle lavoratrici e dei lavoratori; il Mezzogiorno. Sono queste le priorità su cui abbiamo lavorato come sinistra (Partito della Rifondazione Comunista, Sinistra Democratica, PDC e Verdi), insieme al tema della riduzione dei costi impropri della politica, su cui, per brevità, non mi soffermo, in quanto condivido pienamente ciò che hanno detto prima di me i senatori Battaglia e Villone. Si va avanti, insomma, rispetto alla scorsa finanziaria, sul tema del precariato, definendo bene le procedure per la stabilizzazione, i requisiti di anzianità di servizio secondo legge, un programma triennale di fabbisogni e un piano di stabilizzazione per il personale non dirigenziale.

fino alla stabilizzazione devono avere continuità, avremmo rischiato un paradosso. Voglio però soffermarmi brevemente anche su un altro aspetto. Ieri Nicola Rossi sul «Corriere della Sera»

idealmente ai critici come Rossi, ma soprattutto ai senatori di quest'Aula, che è del tutto evidente - basta una lettura del testo - che, prima o dopo, una procedura selettiva o un concorso vi sarà; quindi, non vi è alcun aspetto di illegittimità. La seconda domanda che mi verrebbe da rivolgere a Rossi è la seguente: ma dov'eri, Rossi, quando si assumevano tanti precari nelle pubbliche amministrazioni? Quando nessuno si poneva il problema di come i progetti venivano dilatati? O quando, tagliando le risorse agli enti locali, si tollerava appunto che in maniera impropria si procedesse ad assunzioni che non avevano poi una corrispondenza? Infine, vi rivolgo un'ultima domanda: come avrebbero funzionato in questi anni le pubbliche amministrazioni, senza il ricorso a queste forze? La verità è questa: da una parte, alcune componenti ultraliberiste del Parlamento e delle istituzioni monetarie avevano lavorato per negare ogni possibilità di spesa pubblica finalizzata al risarcimento sociale in questa finanziaria.

una grande mobilitazione: è la manifestazione del 20 ottobre, centrata proprio sui temi della lotta al precariato e per il salario delle lavoratrici e lavoratori, che ha riaperto la discussione, rafforzato l'unità della sinistra e che quindi ci ha permesso per la prima volta di gestire unitariamente sia gli emendamenti sia la scelta delle priorità. Da questo punto di vista, pur non avendo nessuno spazio il trionfalismo, credo dobbiamo essere molto soddisfatti

frutto della continuità nella lotta all'evasione fiscale, a riduzione della pressione fiscale sui lavoratori dipendenti, a partire dalle fasce di reddito più basso, elevando per le aliquote più basse la quota di detrazione per le spese di produzione del reddito. Finalmente, con questo emendamento, la questione salariale del mondo del lavoro dipendente entra in Aula, nelle priorità della maggioranza e del Governo, segnalando una difficoltà specifica dell'Italia nell'Europa. Abbiamo i salari più bassi del 40 per cento rispetto alla media europea e lo dicono tutti, dal movimento sindacale fino ad arrivare al governatore Draghi. Ebbene vorrei garbatamente polemizzare con il collega senatore Ciccanti. Lui dice che non avremmo applicato, prima col decreto, poi con la finanziaria, quanto previsto dal comma 4, articolo 1, della scorsa finanziaria. Non avremmo cioè utilizzato - dice Ciccanti - l'extragettito per ridurre le tasse. Ciò non è vero. Prima col decreto fiscale e prima ancora con il decreto di luglio, con l'aumento delle pensioni minime poi con l'aumento dei fondi sociali, abbiamo inciso sulla condizione dei redditi più bassi contribuendo a ridurre della loro situazione, anche dal punto di vista del prelievo degli incapienti, ma riducendo la povertà, se è vero come è vero che l'ISTAT ha certificato che, seppure in maniera assolutamente insufficiente, queste misure hanno effetto di riduzione della povertà; Ciccanti o chi per lui non volesse dire che la riduzione andava applicata soltanto ai forti e solo alle imprese che pure in questa finanziaria incassano - giustamente, per un verso - allargando la base imponibile, la riduzione dell'IRAP e dell'IRES. credo molto importante che, seppur timidamente - mi rivolgo al collega Viespoli - vi è, con la reintroduzione del credito di imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, finalmente la reintroduzione della priorità Sud nella finanziaria. Sia chiaro: non ci basta che si diano 333 euro per ogni assunto e 416 per ogni lavoratrice. La verità politica è un'altra: dopo anni di neoliberismo, dove nel Sud tutto era *deregulation* urbanistica (i famosi accordi di programma) o precarietà e sottosalario (i famosi contratti d'area), finalmente si apre una stagione centrata sui diritti dei lavoratori, sulla salvaguardia ambientale del territorio, sull'obiettivo di un piano per lo sviluppo e per il lavoro. Ha ragione Viespoli: servirebbero più risorse! Cercheremo nelle prossime settimane e mesi di procurarle a partire da un punto che reputo negativo: il non accoglimento del nostro emendamento sul reddito minimo d'inserimento teso a cofinanziare con 100 milioni le Regioni, non solo del Sud ma anche del Nord come il Friuli, che hanno concretamente avviato l'esperienza di inclusione sociale attraverso un reddito di cittadinanza.

rappresenta un elemento di continuità con la legge contro gli infortuni che quest'Aula ha approvato, anche ascoltando il richiamo delle alte cariche dello Stato.

dei senatori in quest'Aula e anche del significato di grandi lotte sociali per la democrazia e lo sviluppo, credo che il Senato tutto intero debba essere soddisfatto del proprio lavoro.

Vedete, il Ministro dell'economia, aprendo questo dibattito in Aula, ha svolto una considerazione, in parte interessante, in parte contraddittoria.

Anzi, secondo me, con essa si è distrutto anche quel minimo di risorse che i cittadini, nella loro capacità di risparmio, hanno creato in questi ultimi anni.

insieme, di questa manovra finanziaria e di bilancio in qualche modo è contenta. No, sono tutti scontenti. È la prima volta nella storia di questo Paese che c'è uno scontento generale. Non si può dire nemmeno che si chiedono sacrifici oggi per dare benefici domani, perché non ci sono le condizioni. Che significato ha ha poi dire che modifichiamo il tipo di approccio della distribuzione delle risorse, non più basata sul vecchio sistema, che abbiamo utilizzato per tanti anni, ma individuando 34 missioni e circa 180 programmi? Il programma non ha portato buona fortuna a questo Governo; lasciamo stare le missioni, lasciamo stare il programma, cerchiamo di interpretare i bisogni della gente, delle giovani generazioni, delle persone ai margini di questa società,

la pubblica amministrazione. Una volta si diceva che erano i pensionati la causa dei mali del nostro Paese; adesso no, sono la pubblica amministrazione e i fannulloni al suo interno. Vi rendete conto che le risorse stanziate per il 2006 e il 2007 non coprono nemmeno

sono queste le parole utilizzate dal presidente Prodi per definire i documenti della manovra di finanza pubblica per il 2008 all'esame del Parlamento. Il Senato ha già affrontato, con estremo senso di responsabilità, l'esame del decreto collegato, approvato il 25 ottobre scorso, rispettando il calendario dei lavori prefissato. Contestualmente, la Commissione bilancio ha iniziato e concluso giovedì scorso i suoi lavori con l'accoglimento di molte significative modifiche al disegno di legge originario, procedendo ad un confronto serio, anche in questo caso, nei tempi prestabiliti. Oggi l'Aula si trova a discutere, dopo aver superato con grande serenità la prova del voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, un testo, come ho già detto, contenente novità su temi importanti quali il precariato, il sostegno alle famiglie, l'occupazione nel Mezzogiorno. Sul fronte del precariato, l'intesa raggiunta dalla maggioranza ha consentito l'approvazione di un testo che prevede che le amministrazioni pubbliche predispongano, entro il 30 aprile 2008, un piano triennale per la progressiva stabilizzazione del personale precario non dirigente, con uno stanziamento aggiuntivo (per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010) di 20 milioni di euro rispetto ai 5 già previsti. Per quanto riguarda le famiglie, vorrei ricordare alcune previsioni utili ad apportare sollievo ai cittadini gravati oggi più che mai dal caro vita:

lo stanziamento di 30 milioni di euro per rideterminare gli assegni alle famiglie con membri inabili e orfani; ancora, l'eliminazione del tetto di 50.000 euro per usufruire degli sgravi ICI, escludendo dal taglio le ville, le case di lusso e i castelli. Importante, poi, la dotazione di 200 milioni l'anno per i prossimi tre anni per il credito d'imposta per la creazione di nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, con particolare attenzione nei confronti delle donne lavoratrici svantaggiate. Sul fronte sicurezza, è stato introdotto un *bonus*, fino a un massimo di 3.000 euro, a favore dei tabaccai che vorranno istallare telecamere, *bancomat* e sistemi di sicurezza nei propri esercizi commerciali. Infine, vorrei citare gli importanti segnali lanciati da questa maggioranza sul fronte dei tagli ai costi della politica: anzitutto, la riduzione dei membri dell'Esecutivo, che non potrà superare i 60 componenti, e in particolare i titolari dei dicasteri non potranno essere più di 12, così come previsto dalla legge Bassanini del 1999. Poi, i tagli ai costi della politica locale: con la riduzione del numero degli assessori nei grandi enti; con la nuova disciplina dei gettoni di presenza che in nessun caso potranno essere trasformati in indennità e superare come importo mensile il 25 per cento dell'indennità massima del sindaco e del Presidente; con il divieto di aspettativa per i consiglieri comunali e provinciali. Dunque, tagli significativi che serviranno a finanziare misure come l'abolizione dei *ticket* sanitari sulla diagnostica. Non ultimo, voglio ricordare l'approvazione di un emendamento in Commissione bilancio (contenente un errore tecnico che verrà corretto) per ripristinare l'adeguamento dei compensi dei magistrati tagliati dalla finanziaria 2007: una battaglia di giustizia - per dirla con un gioco di parole - volta a sanare una situazione ingiusta nei confronti della magistratura italiana. Ci auguriamo che la mole di emendamenti presentati dall'opposizione in Aula e l'utilizzo di tempi dilatati per la discussione non impediscano il prosieguo di un confronto serio quale quello iniziato fruttuosamente in Commissione per giungere nei tempi prefissati all'approvazione del disegno di legge finanziaria. *(Applausi

Signor Presidente, questa che ci apprestiamo a discutere e poi votare passerà alla storia come la finanziaria delle grandi occasioni perse. A trent'anni dall'istituzione di questa legge abbiamo trascorso almeno gli ultimi dieci a dirci e a sentirci dire che il metodo andava cambiato e che, se non si riusciva a modificare il sistema legislativo, sopprimendo la legge finanziaria e concentrando la manovra annuale nella sola legge di bilancio per tutti quello del professor Monorchio), almeno si doveva comunque tentare un metodo diverso, un approccio diverso e più virtuoso. L'occasione mancata è ancora più grande se pensiamo alla fase sociale che sta attraversando il Paese. La ventata di antipolitica di questi mesi chiedeva, anzi imponeva un cambio di rotta. Il rapporto fra il cittadino e la politica, così in crisi, doveva vedere in questa occasione una prova di maturità. E invece dai grandi annunci si è passati ai piccoli emendamenti; dal rigore alle marchette. L'opposizione ha fatto e sta facendo la sua parte: pochi, ma mirati emendamenti. Ma la maggioranza no

sacrificando il sottosegretario Sartor a fare da comparsa in un film muto. Il Ministro non ha sentito la necessità di farsi vedere neppure quando si è inaugurato il nuovo sistema di autocertificazione sulla copertura finanziaria del famoso emendamento 3.2000, senza la bollinatura della Ragioneria di Stato. Il Paese chiedeva tagli alla politica, alla casta. Noi di AN siamo stati tra quelli che non hanno riottosamente disprezzato e allontanato il "grillismo", banalizzandolo: i nostri emendamenti al taglio dei costi della politica parlavano e parlano chiaro. I tagli tanto annunciati non ci sono stati; addirittura quelli che erano presenti nel testo base sono stati ampiamente modificati e ridotti. Penso solo alla riduzione del 20 del numero dei consiglieri e degli assessori negli enti locali, che avrebbe comportato 250 milioni in meno: ci si è accontentati di abbassare semplicemente il numero degli assessori da 16 a 12.

assolutamente toccato. Non c'è stato nessuno taglio, neanche alla sua ricca dotazione, evidentemente pensando di avere un momento di crisi politica e quindi nel tentativo di guadagnarsi il suo favore nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.

attività varie che fanno capo esclusivamente a ben individuati senatori eletti all'estero. Tuttavia, l'aggravio determinatosi in quell'ultima notte in Commissione, se contiamo le spese impegnate fino al 2010, arriva a quasi 6 miliardi,

Almeno si andasse all'esercizio provvisorio, afferma qualcuno: il rapporto *deficit-*PIL passerebbe dal 2,4 all'1,8 per cento; pertanto, comunque, sarebbe meglio di quanto realizza questa finanziaria. Non parliamo della stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione, che manca di copertura: la norma parla di 20 milioni, la relazione tecnica di 47,3;

i tagli forse si sono visti in un ambito: quello della sicurezza. Stamattina ce l'hanno detto in italiano, molto chiaramente, i poliziotti e i sindacati di Polizia che erano fuori di questo Palazzo a protestare perché chiedono solamente di avere strumenti e mezzi per difendere meglio il Paese e i cittadini. La risposta ce l'hanno data loro: i tagli sono stati fatti. Stiamo attraversando un periodo di *slogan*, di patti per la città e di pacchetti. I nostri emendamenti erano molto mirati in questo senso: un miliardo per la Polizia, per i Carabinieri,

Non dimentichiamo che è stato persino eliminato il fondo di riqualificazione urbana (l'articolo 12, comma 3, è stato soppresso), che tanto beneficio aveva dato ai Comuni, perché la sicurezza parte anche dalla riqualificazione delle città. È stato eliminato anche il fondo non eliminato anche il fondo non solo per i tabaccai, ma per tutti i commercianti, che sono presenza attiva nel territorio per la sicurezza dei cittadini. Poi si donano 150 milioni per rimpinguare il fondo dei Rom. Mi avvio a

Sono quindi gli stessi cittadini che vi chiedono di non mancare all'ultima delle occasioni che avete: l'occasione di poter lasciare il Governo di questo Paese per andarvene a casa.

nell'accingermi ad esprimere il giudizio dei Repubblicani sulla legge finanziaria per il 2008 non posso non partire dalla constatazione che un coro di critiche ha accompagnato il varo di questo provvedimento, senza distinzione fra economisti amici e analisti prevenuti. Contro l'impostazione della manovra hanno infatti parlato uomini come Mario Monti, Tito Boeri, Fabrizio Galimberti, Francesco Giavazzi e Guido Tabelloni, solo per citarne alcuni. Carenza di respiro programmatico, sottovalutazione dei grandi problemi strutturali dell'economia, mancanza di coraggio nell'affrontare gli squilibri finanziari più profondi caratterizzano in realtà il provvedimento al nostro esame. Voglio soltanto citare un dato. Il grafico allegato alla relazione tecnica del disegno di legge per l'attuazione del Protocollo sul *welfare* mostra che la spesa pensionistica crescerà nei prossimi 13 anni di 0,1 punto di PIL ogni anno. Alla fine del periodo, quindi, sarà cresciuta oltre un punto di PIL. Era necessario? Nel 2006, secondo le valutazioni dell'ISTAT, la spesa previdenziale è stata pari al 43 per cento della spesa corrente, al netto dei trasferimenti e degli interessi. Era proprio indispensabile ridurre ulteriormente una vita lavorativa già troppo breve rispetto agli *standard* internazionali? E se a questo dato sommiamo il peso della finanza decentrata, pari al 32,1 alle amministrazioni centrali non resta che il 24,9 per cento del totale. Con queste somme dovremmo fare tutto, dalla sicurezza alla ricerca scientifica, agli investimenti in infrastrutture (pari negli ultimi anni ad appena un punto del PIL). La cosa che più sorprende è che di questi problemi il Governo non mostra consapevolezza. Una finanziaria inadeguata, quindi. Inadeguata di fronte ai problemi, incapace di tracciare una rotta che orienti le grandi scelte collettive verso traguardi in grado di mettere al riparo l'Italia da una crisi, quella internazionale, di cui ancora oggi è difficile valutare la portata e le possibili conseguenze. Scarso coraggio, in definitiva, e poca lungimiranza. Conseguenze inevitabili di una maggioranza divisa su tutto. Immaginiamoci su quelle scelte di fondo che presuppongono un cemento culturale comune e un sistema di valori condiviso. Gli italiani non meritano questa finanziaria. Ci fossimo trovati di fronte ad una irresponsabilità diffusa o al rifiuto del Paese di misurarsi con le sue difficoltà, l'avremmo capito: davanti a fenomeni di rigetto, sarebbe stato giustificato anche un atteggiamento rinunciatario. Ma oggi qual è la situazione? Vi sono forse stati fenomeni di apatia, di indifferenza, di non condivisione nello sforzo di superare la crisi da parte del Paese? Direi proprio di no. Guardiamo ai dati. Il 6 dicembre dello scorso anno, ad un passo dall'approvazione della legge finanziaria, il vice ministro Visco presentò qui in Senato le sue previsioni di entrata. Le calcolò in 33,858 miliardi. Solo pochi mesi dopo, l'ISTAT indicò invece una cifra pari a 46,273 miliardi, con una differenza pari a 12,414 miliardi. Forse, se le previsioni fossero state più accurate, fin da allora si poteva scrivere una finanziaria diversa ed evitare uno *shock* depressivo all'economia italiana. A consuntivo si può dire che il primo tesoretto è stato pari a circa 1,2 punti di PIL, tanto che il *deficit*, previsto dalla Nota di aggiornamento al DPEF nel 3,6 per cento, al netto delle spese *una tantum*, si è ridotto al 2,4 nel frattempo, tuttavia, la pressione fiscale è cresciuta di 1,7 punti e le spese di 1,9. Nel 2007 abbiamo assistito alla stessa sceneggiata: di nuovo le previsioni di entrata sono state sottostimate, di nuovo il miracolo di un tesoretto che nasce come Venere dalla spuma del bilancio. Il totale delle maggiori entrate, accertate in due distinte *tranche*, è stato pari ad oltre 14,5 miliardi di euro. Ve ne sarà un terzo, che spunterà durante la discussione in Aula a Montecitorio, pronto per essere speso su richiesta della sinistra antagonista? Non ne conosciamo l'importo esatto, ma è credibile che l'ordine di grandezza superi i 3 o i 4 miliardi di euro

o non si forniscono le cifre esatte al Parlamento e all'opinione pubblica che assiste sconcertata al susseguirsi delle docce scozzesi, per cui in un momento siamo al 1992, il giorno dopo i conti pubblici sono risanati, grazie all'indefessa azione del Governo. Mi auguro che nella sua replica il Ministro dell'economia possa mettere fine a questo balletto ed assumersi le sue responsabilità. Se i grandi sacrifici degli italiani, che hanno pagato senza battere ciglio più di quanto era stato loro richiesto, fossero stati premiati, oggi il *deficit* sarebbe stato pari all'1,4 nel 2008 sarebbe inferiore all'1 per cento, ad un passo dalla più virtuosa Germania. Queste risorse, invece, sono state sprecate in una politica senza costrutto, fatta di piccole mance e di interventi a pioggia che non hanno recato vantaggio alcuno, non hanno dato reale sollievo alle zone di disagio sociale, non hanno rimesso in moto il processo di sviluppo, visto che l'Italia è all'ultimo posto della classifica europea, non hanno alimentato quel processo di riforme che è indispensabile per superare lo stato di incertezza profonda in cui versa il Paese. Diciamo la verità: quel che manca è l'indicazione di una rotta, per cui gli interventi si sommano e si contraddicono in un gioco a saldo zero, anzi negativo, vista la regressione in atto nei tratti di fondo dell'economia nazionale. Se però manca la rotta, le responsabilità prime sono del Presidente del Consiglio, che per sopravvivere è costretto ad una continua, quanto paralizzante, opera di inconcludente mediazione. Negli scorsi mesi il Partito Repubblicano aveva indirizzato una lettera aperta al Ministro dell'economia: gli avevamo offerto tutto il nostro appoggio su una linea di rigore al servizio dei grandi interessi nazionali. Rinnoviamo la nostra disponibilità, ma che Padoa-Schioppa faccia sul serio il Ministro dell'economia, si faccia forza del suo sapere tecnico da economista qual è, ricorra al linguaggio dei numeri, non replichi con battute che producono effetti controproducenti, e sappia dire di no. I grandi Ministri del tesoro della storia italiana hanno sempre parlato poco ed operato con mano ferma, anche quando le condizioni politiche avrebbero chiesto di largheggiare. Padoa-Schioppa proviene dal vivaio della Banca d'Italia, non dovrei essere dunque io a ricordargli l'insegnamento di Guido Carli, quando Antonio Giolitti, allora Ministro del bilancio, inseguiva il sogno della programmazione, e il Governatore della Banca d'Italia realizzava - era il 1964 la prima stretta creditizia del dopoguerra, perché chi ha la responsabilità delle finanze pubbliche ha una missione da compiere e non può sottostare alle contrastanti pressioni settoriali. Non prometta quindi il Ministro cose che non può mantenere, come l'ipotetico taglio di spese, per un importo pari a 21 miliardi di euro, come indicato nell'ultimo DPEF. Il Paese ha bisogno del linguaggio duro e amaro della verità. Forse usarlo contribuirebbe a far saltare gli equilibri di questa composita maggioranza, ma è meglio che saltino questi equilibri piuttosto che le prospettive di sviluppo del nostro Paese.

colleghi, questa finanziaria, per quanto riguarda i settori dell'istruzione, dell'università e della ricerca appare sicuramente deludente. Inizierò dall'università. È una finanziaria non solo deludente ma che, con riferimento all'università, nasconde anche una sostanziale truffa politico-contabile. Ilministro Mussi e i membri della maggioranza hanno sbandierato - lo abbiamo sentito anche negli interventi

I dati sono 7 miliardi e 87 milioni di euro per il fondo di finanziamento ordinario per il 2007; 6 miliardi 868 milioni di euro per il 2008. Dunque, sono già 220 milioni di euro che devono essere decurtati dai 52. Aggiungo però che i tecnici del tesoro sono stati particolarmente abili perché hanno in qualche modo occultato altri tagli e altre diminuzioni di spesa. Basti pensare, per esempio, che non sono esplicitati finanziamenti al fondo per l'edilizia universitaria come non lo sono i finanziamenti per il diritto allo studio sempre previsti in passato, ma in quell'equivoca formulazione che si coglie al comma 1, dell'articolo 52, si dice che che questi 550 milioni di euro sono destinati a finanziare un fondo, che finanzierà a sua volta il fondo di finanziamento ordinario, e che servirà per finanziare, per la parte residua, le spese correnti e quelle diinvestimento

Negativo appare anche l'articolo 92, in particolare con riferimento all'università e alla ricerca. Con riferimento a questo articolo, che come ben si sa

in rapporto con gli altri Paesi OCSE per i quali la carriera di ingresso è flessibile, ma soprattutto perché introduce rigidità molto gravi e fortemente penalizzanti sotto il profilo economico per quanto riguarda l'utilizzo del personale non docente. Non vi è nulla per i ricercatori e i dottorandi di ricerca. Cari colleghi, un dottorando di ricerca prende 800 euro al mese: voi pensate veramente che i ragazzi più bravi vogliano intraprendere una carriera difficile come quella universitaria, quando la prospettiva è di guadagnare, a 26 anni, 800 euro netti al mese? al mese? Il ministro Mussi si era dichiarato disponibile ad appoggiare un nostro emendamento, che prevedeva un aumento di 40 milioni di euro per pagare di più i dottorandi di ricerca. Noi proponiamo anche un incremento significativo dei fondi, in particolare del fondo di finanziamento ordinario, tenendo conto che vi sono 15 miliardi di extragettito che non sono stati utilizzati, che vi sono 3 miliardi e mezzo di spese clientelari destinate ai vari Ministeri, e che addirittura ribadite l'assegno di mantenimento per i Rom: credo che il nostro sia l'unico Paese al mondo che prevede una misura di questo tipo!

finanziaria) secondo percentuali ben precise. È la prima volta che si propone - e credo sia un passaggio molto importante - che più della metà degli investimenti sia destinata per la valorizzazione dei docenti più bravi, per il diritto allo studio, per l'edilizia universitaria e, soprattutto, per il riequilibrio a favore delle università virtuose. Se ne parla tanto, ma poi alla resa dei conti non si fa nulla al riguardo. Penso anche che si debba eliminare l'articolo 92, in particolare per quanto riguarda le università e gli enti di ricerca, perché costituisce indubbiamente un elemento senz'altro penalizzante.

e in parte ha peggiorato le riforme varate dal centro-destra nella scorsa legislatura. In questa finanziaria, certamente viene peggiorato quanto fatto da noi. Uno dei passaggi più importanti della legge n. 53 del 2003 era la riforma del reclutamento, che finalmente ci metteva al passo con le migliori esperienze europee. Penso per esempio a quella della Finlandia. Prevedevamo infatti il numero programmato per l'accesso al biennio specialistico universitario, il tirocinio,

gli organici di diritto, ma ne avete tagliati 30.000 sugli organici di fatto. Non ci sono soldi per i contratti per il personale, anzi, addirittura le risorse sono inadeguate per il pagamento della vacanza contrattuale. Date per scontato che per un anno, come già avete fatto quest'anno, non pagherete gli aumenti di stipendio. Non si prevede nulla per la valutazione delle scuole e per l'assunzione dei precari. Avete preso in giro 100.000 persone che non vedono alcun finanziamento al riguardo. Chiedo veramente un'inversione di rotta. Abbiamo presentato emendamenti per pagare di più gli insegnanti più bravi, per tutelare i docenti e soprattutto per garantire i ragazzi disabili, offrendo loro opportunità con insegnanti di sostegno

onorevoli membri del Governo, colleghi senatori, Joaquin Almunia, commissario dell'Unione Europea agli affari economici e monetari ha bollato la finanziaria italiana per il 2008 come «poco ambiziosa». Non poteva essere altrimenti dopo la finanziaria 2007 e da allora 12 mesi di Governo Prodi che hanno acuito nel Paese lo scontro sociale l'insicurezza, la recessione e la sfiducia totale nelle istituzioni fino ad arrivare al trionfo dell'antipolitica. Questa finanziaria, che più modestamente definirei del «tirare a campare», sembra più preoccuparsi dell'effettiva sopravvivenza del Governo, attraverso interventi diffusi e poco significativi, che ricercare un'impostazione fortemente selettiva quale presupposto necessario a una politica riformista e poco incline alla deriva. Come nelle 280 pagine del programma elettorale, questa maggioranza continua a non decidere e a non cambiare, esercitandosi in un tiro alla fune che poche volte ha registrato un coraggioso strappo verso una coesa ed univoca volontà di prendere le redini del Paese, anziché esercitare il potere direi fine a se stesso senza una solida progettualità. È ciò che il cittadino percepisce ed è ciò che alimenta l'odio verso la casta. Questo vale naturalmente anche per il comparto agricolo, che deve registrare ancor prima di introdurci in un dettagliato esame della finanziaria 2008, la mancata attuazione di quanto previsto dalla finanziaria dello scorso anno. Le promesse del 2007 con 977 milioni di euro sono state, a dispetto delle attese, per la gran parte disattese. I provvedimenti sulle crisi di mercato e sul credito d'imposta per l'internazionalizzazione delle imprese sono ancora all'esame della Commissione europea. Gruppi di lavoro ministeriali stanno ancora scrivendo i piani forestali e i piani di settore. I decreti attuativi del Fondo per la competitività e lo sviluppo sono in istruttoria. L'attuazione del comma 382 dell'articolo 1 della finanziaria 2007 sulle agroenergie trova attuazione nel decreto di accompagnamento alla finanziaria che stiamo esaminando, ed è stato votato pochi giorni fa grazie anche a un forte impegno di Alleanza Nazionale. Potremmo fare molti altri esempi, ma è evidente che la poca autorevolezza a Bruxelles e le grandi difficoltà del Governo Prodi alla concertazione interministeriale compromettono la progettualità del lungo periodo con un'insanabile discrasia tra impegno e relativa realizzazione. Il presidente della Coldiretti, dottor Sergio Marini, davanti al ministro De Castro ha così concluso il suo intervento al 7° Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione del 19 e 20 ottobre scorso: «potete solo migliorare» e «se proprio dovete fare qualcosa cercate di stare fermi, fate lavorare solo le imprese». Sono parole pesanti come macigni, quelle degli agricoltori, dopo una luna di miele durata poco e che rischia di trasformarsi con questa finanziaria in un vero e proprio divorzio. In Italia tutti gli agricoltori stanno vivendo una spaventosa crisi di liquidità derivante da emergenze fitosanitarie alle quali non sono corrisposti indennizzi da parte dello Stato, che è in ritardo anche con i pagamenti di tante calamità. Registriamo dei ritardi anche nel saldo dei premi PAC da parte dell'AGEA, che eroga con la velocità del bradipo e spesso si dimena tra errori e complessi meccanismi di verifica. Il rallentamento generale dei bandi regionali dei Piani di sviluppo rurale, il costo della mano d'opera alle stelle anche a causa di oneri previdenziali insostenibili, così come il generale aumento dei costi alla produzione completano il quadro. Il cambiamento climatico e la continua oscillazione dei prezzi tra produzione e dettaglio rendono l'agricoltore il soggetto debole della filiera. In questa poco rosea prospettiva, Alleanza Nazionale ha avanzato richieste precise in questa finanziaria, in minima parte accolte dalla Commissione agricoltura prima e dalla Commissione stabilizzazione fiscale del comparto agricolo ed estensione del regime agevolato anche alla pesca; integrazione dello stanziamento a favore del settore bieticolo-saccarifero; realizzazione di un secondo piano irriguo per far fronte a siccità e dissesto idrogeologico; stanziamento di risorse per il Corpo forestale dello Stato, chiamato a far fronte come non mai alla emergenza incendi; potenziamento e razionalizzazione del sistema dei controlli per il settore agricolo e agroalimentare; incremento del Fondo per la montagna (rivedendo l'esclusivo criterio altimetrico per la definizione delle Comunità montane con maggiore attenzione al sistema complessivo che tenga conto della denatalità, dell'invecchiamento della popolazione grazie a tutto introduzione di un serio sistema di monitoraggio e controllo dei prezzi lungo l'intera filiera a tutela, da una parte, dei produttori e, dall'altra, dei consumatori; esenzione dell'imposta di bollo per tutti gli atti inerenti la formazione, l'accorpamento o l'arrotondamento della proprietà coltivatrice; esenzione da accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra ed istituzione di un fondo per l'adeguamento dei processi produttivi delle aziende zootecniche relativamente all'inquinamento provocato dai nitrati. Questi sono alcuni degli interventi richiesti da Alleanza Nazionale la cui analisi delinea il quadro e lo stato di salute dell'agricoltura italiana della quale troppo poco si discute nelle Aule parlamentari e solitamente in circostanze di emergenza quali calamità ed epidemie. La realtà è quella di un comparto che quest'anno, dopo una positiva tendenza fino al mese di marzo, ha visto nuovamente ridursi il reddito, dovendo fare i conti, peraltro, con una insensata campagna stampa contro l'aumento dei prezzi al consumo del quale gli agricoltori sono stati ingiustamente ritenuti responsabili. Proprio nel corso dell'indagine conoscitiva della Commissione agricoltura del Senato è emerso il ruolo antinflattivo svolto nel passato dalla agricoltura italiana a causa della scarsissima dinamica dei prezzi all'origine. Ora sono cause congiunturali internazionali, come gli eventi climatici per i cereali, o strutturali, come l'esaurimento degli *stock* ed in generale l'aumento della domanda dalle economie emergenti verso sbocchi alternativi, quali i biocarburanti, a condizionare i prezzi in Italia. In questo quadro il presidente della Confagricoltura, dottor Vecchioni, chiede una nuova «politica per le *commodities* in Italia e uno slancio nuovo per esaltare a Bruxelles le politiche agricole nazionali e non per omologarle: altrimenti l'Italia sarà più debole e vincerà il più forte». Alleanza Nazionale crede profondamente nel tratto identitario dell'agricoltura italiana non assimilabile ad altra in Europa e per questo nella necessità di serie politiche di controllo sulla qualità e sulla contraffazione dei marchi e sulla tutela del valore sociale e culturale della sana alimentazione italiana. La tanto declamata multifunzionalità dell'agricoltura non trova applicazione nelle previsioni di questa finanziaria né in materia di assetto del territorio (abbiamo sottolineato con un emendamento la necessità di mantenere un ruolo attivo ai consorzi di bonifica e agli agricoltori nella prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi) né in materia di riduzione della filiera. Non è vero, io credo, che tutte le battaglie per l'agricoltura si conducono a Bruxelles. Certo dovremmo vigilare che la prossima riforma dell'OCM vino non produca effetti devastanti con estirpazioni ingiustificate e poche garanzie per la qualità italiana con l'ammissibilità dello zuccheraggio e l'etichettatura secondo sistemi non rispettosi della qualità. Ma da oggi al 2013, quando cesserà il regime delle quote, come ci ha chiarito proprio qui in Senato la commissaria europea Fischer Boel, dovremo aver fatto qualcosa per la salute e la competitività delle aziende agricole italiane. Il problema del costo del lavoro rimane un punto centrale in agricoltura sul quale attendiamo di verificare il protocollo sul *welfare* che promette riduzione della pressione INAIL e possibilità di lavoro accessorio. Ma anche la ricomposizione fondiaria e la semplificazione amministrativa, l'accesso al credito e meccanismi stabilizzatori dei prezzi sono per l'agricoltura la premessa per sostenere la sfida del mercato globalizzato, ma anche la politica aggressiva dei vecchi e nuovi *partners* dell'Unione Europea. Attualmente l'Unione Europea ha solo 5.000 tonnellate di riserva di grano. Non accadeva da tempo immemore. Un fatto ignorato da molti ma che dovrebbe farci riflettere, invece su possibili, futuri, sconfortanti scenari. Una riflessione seria, e concludo, che renda al settore primario la sua «primarietà».

Ma anche perché si raccolgono i primi frutti dell'avvio del processo di riforma della sessione di bilancio, promosso dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato, insieme al Governo. Come ha ben illustrato il senatore Albonetti, con il nuovo sistema di classificazione per missioni e programmi, il bilancio dello Stato è diventato finalmente più leggibile e trasparente, rendendo comprensibile anche ai non esperti come si distribuiscono le risorse finanziarie disponibili sulla base delle leggi già esistenti. È un primo passaggio, fortemente voluto dal ministro Padoa-Schioppa, che può contribuire non poco, in futuro, a migliorare i termini del dibattito sulla cosa pubblica, spostando l'attenzione da "chi" gestisce a "cosa si fa" con le risorse. Da questo passaggio, si è anche inteso come sia fuorviante, da parte del Parlamento, concentrarsi solo sulla legge finanziaria, cioè sulle variazioni marginali apportate ogni anno (che in questo caso incidono Per incidere sulla qualità e sulla quantità della spesa pubblica è necessario porre al centro dell'attenzione l'intero bilancio, i criteri di allocazione e le modalità di utilizzo dell'insieme delle risorse pubbliche, superando la logica dell'approccio incrementale (responsabile, non in piccola misura, della tendenza all'aumento continuo della spesa e della sua scarsa qualità). Certo, sono necessari ulteriori passi per aumentare la coerenza tra programmi e strutture amministrative e per rendere la gestione della spesa pubblica maggiormente flessibile e orientata ai risultati. Per questo incitiamo il Governo, e il Ministro dell'economia in particolare, a continuare con determinazione su questo percorso, che richiede tempo, ma che è necessario affrontare, se si vuole contenere la spesa e, al contempo, migliorare la qualità dei servizi offerti dalle A tal fine, sarà opportuno concordare quanto prima, tra Governo e Parlamento, l'elaborazione di indicatori di *performance* delle attività delle pubbliche amministrazioni, per mezzo dei quali si potrà accertare non solo "cosa si fa" con le risorse (obiettivo ormai raggiunto), ma anche "come lo si fa". Quanto al merito della manovra, mi limito a poche e brevi riflessioni, per evidenziare come la bontà di un impianto che punta ai tre grandi obiettivi del risanamento, dello sviluppo e dell'equità vada ulteriormente migliorata tramite una maggiore capacità selettiva degli interventi. La manovra, nel suo complesso, opera una parziale restituzione dell'extragettito: ne beneficiano le famiglie, in particolare incapienti e proprietari di prima casa, oltre ai conduttori di immobili sotto ad un certo limite di reddito. Va sottolineato, per inciso, come si tratti di misure che danno attuazione al disposto del comma 4, dell'articolo 1, della legge finanziaria approvata l'anno scorso. Ciò, tra l'altro, avvalora quanto dichiarato dal senatore Legnini circa la portata normativa - quindi vincolante, non meramente programmatica della disposizione inserita anche quest'anno al comma 4 del disegno di legge finanziaria: si tratta dell'impegno ad utilizzare prioritariamente l'eventuale ulteriore extragettito nel 2008 alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti. Sicuramente positivi sono gli effetti redistributivi delle misure a favore degli incapienti, che hanno il pregio di dare sostegno a quei soggetti sino a qui sempre esclusi, per definizione, da ogni tipo di agevolazione fiscale. Si tratta di benefici che, per agire in senso veramente redistributivo, dovrebbero essere resi strutturali, mentre si è preferito dare carattere di beneficio permanente alla riduzione dell'ICI. Una scelta che, anche se risponde ad un'istanza sociale sentita e diffusa, nelle modalità attuative rischia di essere discutibile e costosa; forse, avrebbe potuto lasciare il posto a provvedimenti di sgravio fiscale e di spesa a sostegno delle famiglie, partendo dalle fasce di reddito più basse. Invece, la misura in oggetto, così com'è concepita, rischia di dare un'agevolazione - maggiore in valore assoluto, ma uguale in percentuale - a chi ha rendite della prima casa più elevate perché vive in Comuni più grandi o a maggior tensione abitativa; potrebbe inoltre risultare più generosa nei confronti dei contribuenti con reddito medio-alto. Se poi si considera che l'ICI rappresenta il principale tributo proprio dei Comuni e che costituisce circa il 24 per cento delle loro entrate correnti, non appare opportuna una sua riduzione decisa a livello centrale e compensata con trasferimenti statali, dunque con ulteriore finanza derivata, finanza derivata, in contraddizione con l'impegno ad attuare finalmente il federalismo fiscale. Pertanto, ci auguriamo che, proprio nell'ambito del percorso parlamentare di attuazione del Titolo V della Costituzione, si possa passare da misure poco selettive, come questa, ad una più funzionale distribuzione delle risorse tra i livelli di Governo territoriali, che consenta ai Comuni stessi di rafforzare ulteriormente, nell'ambito della loro autonomia e con un'azione più incisiva ed efficace, le misure agevolative sulla prima casa, già poste in essere dalla gran parte degli enti locali. Di rilievo sono anche gli interventi destinati dalla manovra allo sviluppo. Ricordo, solo per citare qualche esempio, gli interventi fiscali per società ed imprese. Si preannunciano a costo zero ma potranno avere effetti significativi sia sulla competitività che sulla ripartizione del carico fiscale tra i diversi soggetti. Un aspetto di particolare importanza è anche l'impegno a semplificare e rendere più certe nel tempo le norme fiscali. Rilevanti anche le misure per le piccole imprese. La finanziaria rivoluziona su base volontaria il trattamento fiscale di un insieme molto ampio di lavoratori autonomi e piccole imprese. Si tratta di un intervento a costo quasi nullo per l'erario, ma che ha la funzione di semplificare gli adempimenti fiscali di questi soggetti, riducendone sensibilmente i costi. Infine, una parte rilevante dell'extragettito, destinata allo sviluppo, è andata a rimpinguare le spese in conto capitale, in particolare quelle infrastrutturali, mentre 5 miliardi, poco meno di un terzo dell'extragettito, sono destinati a ridurre l'indebitamento. Non possiamo non riconoscere che l'avvio del risanamento intrapreso con forza e determinazione da questo Governo, lungi ancora dall'essere conseguito, appare rallentato pur nel rispetto degli impegni assunti in sede europea e sia pure per ragioni politicamente comprensibili e persino giustificabili. Dobbiamo tuttavia essere consapevoli che il risanamento, proprio perché non può fondarsi su un ulteriore aumento delle entrate, passa necessariamente per una maggiore capacità di riqualificazione e riduzione della spesa pubblica: principio peraltro tenuto fermo in questa manovra, che ha visto in Commissione un notevole sforzo di ricerca di coperture alternative all'aumento delle pressione fiscale, quali ad esempio la significativa riduzione di alcuni costi della politica. Se molto dunque è stato fatto in un tempo relativamente limitato, l'attenzione e lo sforzo risanatori non vanno tuttavia allentati. Ci aspettiamo che dall'approvazione di questa manovra tragga rilancio l'azione di buon Governo di questo Paese, che ha bisogno anche di una maggiore capacità di confronto costruttivo tra maggioranza ed opposizione sui grandi temi e le riforme di cui ha bisogno il Paese, a cominciare appunto dalle riforme necessarie a perseguire in modo più efficace quella emergenza nazionale, che è il risanamento dei conti pubblici. Ciò richiede la consapevolezza da parte del Parlamento, che sviluppo ed equità passano attraverso una maggiore capacità selettiva delle priorità dell'azione pubblica e la generale condivisione, anche in questa Aula, che lo strumento della legge finanziaria deve essere il luogo del confronto sui grandi temi della politica economica del Paese e non l'atto deputato a risolvere le molteplici istanze di produzione legislativa, tanto meno a soddisfare quelle meramente localistiche.

onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, la finanziaria, così come modificata dal prezioso ed intenso lavoro della Commissione bilancio, completa ed integra il decreto-legge fiscale e prosegue con forza nell'impostazione che collettivamente ci siamo dati sul risanamento, misure di redistribuzione sociale e innovazione ambientale: i tre assi su cui si è mosso il Documento di la missione dell'intera manovra per il 2008, che finalmente quest'anno - lo voglio dire con chiarezza - comincia ad avere ed a fare intravedere un suo progetto, appunto una sua missione. Un primo segnale di redistribuzione si era già avuto con il decreto n. 81 sulle pensioni minime (0,4 punti di PIL). Lotta all'evasione, recupero di base imponibile e restituzione progressiva ai contribuenti

Nella manovra di quest'anno si procede in questa direzione con l'utilizzo dell'extragettito nel decreto fiscale per gli incapienti, come previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della scorsa finanziaria finanziaria ed altre misure sociali. E' già indicata per il prossimo anno la collocazione del recupero di nuove risorse dalla lotta all'evasione fiscale proprio nel *fiscal drag* e nella riduzione della pressione verso i lavoratori dipendenti, oggi che, finalmente, la questione dei bassi salari è diventata oggetto di discussione e di riflessione. Significativi sul fronte sociale sono proprio gli interventi, finanziati in parte con tagli consistenti ai costi della politica, per eliminare, ad esempio, il *ticket* sulla diagnostica. È significativa la riduzione dell'ICI sulla prima casa e la detrazione IRPEF

- lo dico anche a coloro che magari interverranno contro questa norma - che qui non si sta parlando di una sanatoria *tout

Dobbiamo riflettere sulla circostanza che l'amministrazione pubblica in questi anni non ha fatto altro, purtroppo, che incentivare l'utilizzo del lavoro precario. Quindi, questa norma, in qualche modo, indica la indica la strada di un piano triennale, ma anche l'obiettivo, fatta questa operazione, di mettere uno stop al ricorso a quella forma di lavoro all'interno della pubblica amministrazione.

di dequalificazione. Serve per puntare a riorganizzare la pubblica amministrazione e a dare finalmente certezza al diritto. Non significa escludere chi ha merito, perché i concorsi si faranno; vi è una riserva del 40 per cento per il tempo determinato e

andiamo piano. Nel DPEF avevamo indicato delle misure; stiamo semplicemente tentando di recuperare con alcune norme il tempo perduto rispetto ad altri Paesi europei. Si è fatta una grande esagerazione in questi giorni. Addirittura, il quotidiano «Italia Oggi» scrive oggi che i Verdi hanno sbancato Prodi, come se avessimo portato a casa chissà quali risorse e quali emendamenti. In realtà (e mi spiace

da fonti rinnovabili, di stanziare 400 milioni di euro per i certificati verdi e circa 1,4 miliardi di euro per il sistema di conto energia, che si sommano a quanto già incentivato per le fonti rinnovabili dal CIP6 e dai vecchi certificati verdi.

nessuno parla), a firma del relatore Legnini, che prevede una riduzione sulle bollette di 600 milioni di euro, proprio per la norma che permette la riparametrazione del costo evitato

alle fonti rinnovabili e abbiamo consentito all'Italia di riprendere un percorso insieme con il resto dei Paesi europei. Vorrei ricordare che abbiamo subìto procedure di infrazione per il modo in cui applicavamo il CIP6 per le fonti assimilate.

è la finanziaria dell'Italietta; dell'Italietta che avete in mente, dell'Italietta piccola piccola, dell'Italietta più povera. Signor Ministro, i dati sono evidenti: un indebitamento netto derivante dalla manovra di 6,5 miliardi di euro, 0,4 punti del PIL, risorse recuperate per 5,4 miliardi, aumenti di spese e sgravi fiscali per quasi 12 miliardi di euro. Una bella torta, su cui ognuno ha messo le sue bandierine; bandierine di partito, per carità, importanti, ma senza futuro. È un'Italietta meno sicura, un'Italietta dove non si destina se non qualche centesimo, per la famiglia; un'Italietta da mangiare. Siamo tornati all'Italietta della politica come costo. L'ultima notte

l'Ulivo 404 milioni; la Sinistra Democratica 51 milioni; il Gruppo per le Autonomie, non parliamone neanche: si tengono le tasse in Sud Tirolo e poi fanno pagare a noi i vari palazzi e gli uffici di giustizia. Ma i voti i voti si devono pagare, signor Ministro, e lei li ha pagati abbondantemente. Ha pagato, per esempio, con i supposti tagli alla Presidenza della Repubblica e alla Corte costituzionale; dove sono andati questi soldi, soldi importanti, derivanti dai tagli ai costi della politica? Sono andati, Presidente, agli italiani eletti all'estero: avevamo giustamente bisogno di avere cinque *pasdaran* venuti da fuori, perché non eravamo capaci di portare via i soldi da soli. Non ci bastavano i Cirino Pomicino e gli altri, persone che che noi rimpiangiamo, perché avevano una cultura politica (la prima Repubblica aveva da insegnarci in questo senso)? No: abbiamo gli italiani eletti all'estero, che vengono giù di notte e prendono 18 milioni di euro; da distribuire come? A chi ha bisogno. In più, il Governo gliene dà altri 14 e altri 4 sono in tabella. Questi sono i soldi che i contribuenti spendono per mantenere la classe politica. Noi ne avremmo spesi in passato, ma questa volta li avete

Poi venite a fare il Partito Democratico a Milano e dite che avete attenzione per il Nord. Lasciateci in pace, non venite più a Milano. Lasciateci lavorare in pace, non occupatevi più del Nord,

Le imprese le avete tassate: avete ridotto in qualche modo l'IRES e l'IRAP, ma avete aumentato la base imponibile e soprattutto andate a colpire chi ha investito.

Presidente, che abbiamo da fare le nostre rimostranze. Questo Paese non fa figli perché non ha un clima di fiducia e un assetto valoriale importante: non sappiamo, cioè, trasmettere la fiducia e la bellezza della famiglia.

che questa finanziaria non raggiunga gli obiettivi necessari sempre, ma in modo particolare vista l'attuale situazione economica e sociale del nostro Paese (cioè la riduzione del debito, il rilancio dell'economia, una maggior giustizia sociale), non lo sostiene solamente in modo convinto tutta l'opposizione;

contenga misure contrarie ai principi importanti dello Stato di diritto o della valorizzazione del merito, come sono le misure sulla regolarizzazione dei precari nella pubblica amministrazione, lo dicono autorevoli esponenti della maggioranza. Che vi siano delle previsioni di spesa non coperte con chiarezza lo dicono in tanti. Dunque, veramente una finanziaria tra le peggiori. Un insieme di misure scoordinate per raccogliere consenso, che dimostra non solo, per l'ennesima volta, le divisioni della maggioranza, ma direi di più: dimostra come questa maggioranza, avendo ormai la consapevolezza di essere giunta ad un punto morto ha messo da parte i disegni di programmazione e fa solo una finanziaria elettorale. Anche le norme che riguardano l'agricoltura ci lasciano insoddisfatti e confermano questo giudizio generale. Poi tutti affermiamo, ed è vero, l'importanza del settore primario; diciamo che questo settore ha bisogno di un forte sforzo di modernizzazione per affrontare i nuovi problemi della globalizzazione dei mercati e sappiamo che l'agricoltura attraversa un momento difficile anche per gli sviluppi della normativa europea. Ebbene, di fronte a questa necessità, cosa avviene? Avviene non solo che non vengono applicate o vengono applicate in modo parziale e con ritardo le norme già approvate nel passato, perché questa finanziaria contiene veramente molto poco, pochissimo e il contenuto che c'è è assolutamente insufficiente. Ad esempio, le agevolazioni fiscali sono solo conferme temporanee e non sono stabilizzate. Certi stanziamenti - mi riferisco, ad esempio, al comparto saccarifero, alla montagna erano poco più che simbolici e sono aumentati di molto poco dopo il lavoro in Commissione; tante voci - si tratta di voci che contano, come gli incentivi per la pesca, la valorizzazione dei prodotti tipici, la repressione frodi - sono state ridotte: ripeto, ridotte. Tant'è che lo stesso parere dato dalla Commissione agricoltura è stato approvato fra il disagio anche dei membri della maggioranza con ben 13 pesanti osservazioni. Stupisce questa condizione? Direi di no, non ci deve stupire troppo, perché continua a perpetuarsi questo atteggiamento del Ministro, della maggioranza e del Governo di disattenzione, di sottovalutazione della nostra agricoltura, che è anche un arretramento pesante rispetto a quanto era stato fatto dal precedente Governo nella scorsa Cito alcuni esempi che confermano questa mia affermazione. Il primo è la critica svolta dalla Coldiretti in modo pesante, direi plateale. Ecco, questa, la maggiore delle organizzazioni professionali del mondo agricolo e che è stata tradizionalmente governativa, ha dato un giudizio che dovrebbe veramente far pensare.

su un problema che non direi fondamentale, cioè l'uso dei trucioli nel processo di invecchiamento del vino. Il terzo (voglio dirlo con forza) è l'atteggiamento del Ministero e della maggioranza verso il problema del vino, che non solo una scarsa incidenza sul processo della nuova OCM vino se è vero, come è vero, che verrà approvata una nuova norma sull'etichettatura che danneggia pesantemente, anzi rischia di scardinare l'impianto forte della nostra viticoltura. Permettere che si facciano etichette con l'indicazione dell'annata per i vini da tavola significa rompere alla base la piramide delle DOC e delle DOCG che - ripeto - è stata importantissima per il progresso di qualità nella nostra viniviticoltura e che permette ad essa di vincere la concorrenza contro produzioni straniere sempre più agguerrite, che riescono a fare qualità a prezzi inferiori, per motivi strutturali e di legislazione. Possiamo vincere questa battaglia solo se continuiamo a percorrere la strada della tipicizzazione, della individualità dei vini, dei collegamenti sul territorio. Questa norma, che sembra piccola, dà un colpo tremendo a questo impianto. In secondo luogo, pur nella sacrosanta

che lo stesso presidente Bertinotti ha definito malata, non può che essere pesantemente negativo.

rispetto agli anni passati in termini di emendamenti presentati e posti all'attenzione dell'Aula.

ma anche con grande senso di responsabilità, tant'è che siamo arrivati in Aula con il mandato al relatore. Allora, non è non è accettabile e non può passare sotto silenzio che un Ministro per i rapporti con il Parlamento minacci da parte del Governo di apporre la questione di fiducia

Cari signori del Governo, è inutile arrampicarsi sugli specchi: se non siete in grado di tenere compatta la vostra maggioranza sui vostri testi e volete apporre il voto di fiducia,

Allora, è inutile continuare ad accusare noi di praticare l'ostruzionismo, perché francamente quella del lupo e dell'agnello è una storiella antica, che spero anche le nuove generazioni di italiani potranno essere poste in condizione di conoscere. La seconda premessa, signor Presidente,

Non è un fatto specifico, di un singolo emendamento, ma una questione di una gravità istituzionale inusitata. Ricordo brevemente la domanda posta al Governo e al Ministro dell'economia. Il Parlamento e l'opinione pubblica italiana devono sapere perché all'emendamento 3.1000 il Governo ha fatto accompagnare la relazione tecnica firmata dalla Ragioneria generale dello Stato

Non c'è un precedente in questi termini, altrimenti saremmo arrivati all'autocertificazione. Se il ministro dell'interno Amato avesse presentato un emendamento chiedendo una maggiore spesa per la sicurezza, sul quale tutti avremmo convenuto, con una stima del Ministero dell'interno di 100 euro e magari una stima della Ragioneria Generale dello Stato di 1 miliardo di euro, quale delle due relazioni tecniche noi, in quest'Aula, avremmo dovuto considerare ai fini della copertura?

di movimentazione di risorse pari a 27,7 miliardi di euro. Questa è la manovra che stiamo discutendo, altro che manovra *soft.* In queste settimane, nei prossimi giorni, manovreremo 27,7 miliardi di euro più la lievitazione che è avvenuta in gran parte quando l'opposizione, per protesta contro la mancata relazione tecnica della Ragioneria dello Stato, è uscita dall'Aula della Commissione bilancio.

quasi automaticamente, un punto in meno di crescita economica e mezzo punto in più di *deficit* pubblico? I numeri di cui stiamo discutendo in quest'Aula, signor Presidente, quelli che risultavano a fine settembre, sono già radicalmente modificati. Avrei potuto capire la posizione del Governo, che dopo avere effettuato una manovra da 42 miliardi, l'anno scorso, si è ritrovato in cascina 25 miliardi di extragettito

Allora, il Governo spieghi cosa intende quando parla di risanamento. Il risultato è che, grazie all'azione di questo Governo, dopo avere nascosto il gettito e le entrate, si è speso l'extragettito in eccedenza rispetto agli andamenti tendenziali del *deficit* pubblico a legislazione vigente, il che vuol dire automaticamente che, con la legislazione prodotta da questo Governo,

Non basta dire che saremo comunque sotto i parametri concordati con l'Unione europea. Con tutto il rispetto per l'Unione Europea, esiste l'articolo 81 della Costituzione italiana, che questo Governo sembra avere abrogato, nel silenzio dell'Aula e anche dell'opinione pubblica.

se il Governo avesse avuto un progetto strategico di politica economica, considerando che l'anno scorso ha movimentato 42 miliardi di euro e quest'anno 27 miliardi

sulla forma di copertura. Noi avremmo preferito infatti che questa fosse ottenuta attraverso i tagli agli sprechi della spesa pubblica, mentre il Governo - come ha fatto - avrebbe potuto proporre di coprirla con aumenti di pressione fiscale. Ma non c'è neanche questo, signor Presidente.

finanziaria disperde 12 miliardi di euro di risorse movimentate in ben 78 voci di spesa. Cari colleghi della maggioranza, l'assenza del progetto strategico di politica economica è palese; basta mettere il in fila i numeri. Ciò che però voi volete nascondere è la presenza di un progetto politico, non di politica economica, perché dietro ad ogni fettina di spesa pubblica dispersa a pioggia, c'è il nome e il cognome di un partito, di una componente, di una specifica rappresentanza della vostra variegata maggioranza. Vi è allora assenza totale di un progetto di politica economica sull'altare della presenza di un preciso progetto politico di distribuzione e di acquisto politico di voti all'interno della maggioranza con i soldi dei cittadini. Qualcuno di voi ha accusato la controparte di comprare dei senatori, cosa tutta da dimostrare e assolutamente ridicola e risibile. Ammesso però che così fosse, almeno in quel caso si sarebbero usati i soldi personali e non quelli dei contribuenti italiani. Chiudo con un'ultima notazione, Presidente. Cari colleghi della maggioranza, vi rendete conto che con 27,7 miliardi di risorse che avete così disperso in due decreti tesoretto e in questa finanziaria, avreste potuto proporre per le famiglie il raddoppio delle detrazioni per i figli per 7 miliardi, l'azzeramento dell'ICI sulla prima casa per 2 miliardi, la deduzione delle spese per l'istruzione dei figli e la deduzione delle spese per gli anziani? Avreste potuto proporre l'azzeramento nell'ambito IRAP per tutte le piccole e medie imprese del monte salari come base imponibile, con la stessa cifra. Avreste potuto proporre un pacchetto sicurezza serio, con almeno 1 miliardo di euro di risorse. Avreste potuto proporre questi cinque o sei temi per la famiglia, per le imprese, per la ricerca, per le infrastrutture e per la sicurezza. In quel caso noi avremmo potuto criticarvi, perché li avreste coperti con maggiori tasse, ma avremmo potuto pure acconsentire su questi obiettivi strategici. La verità

dobbiamo dare atto alla buona volontà del Ministro dell'economia che ha pensato di tornare alle origini, in applicazione esclusiva e precipua dell'articolo 81 della Costituzione, che agli albori della Repubblica vedeva un bilancio che non aveva bisogno di una legge finanziaria che, evidentemente, tenta di risolvere, al momento dell'approvazione del bilancio dello Stato, le istanze e le aspettative della gente, via via crescenti in funzione del divenire dei bisogni del Paese. Ella, Ministro, ha fatto del suo meglio, ma - ahimè - non poteva fare di più, poiché la sua maggioranza è così diversificata e così negativamente articolata in funzione dei piani e dei progetti di ogni singolo partito, divaricata rispetto all'orientamento che deve avere un Governo, che deve essere unico ed univoco, che evidentemente ogni sua buona intenzione non ha sortito il risultato sperato. Questo Paese, signor Ministro, lei lo sa meglio di me, abbisogna innanzitutto di riservare attenzione delle aree deboli del Paese, intendendo per aree deboli quelle laddove vi sono sacche notevoli di disoccupazione, prima tra tutte il Mezzogiorno, e quindi al riequilibrio territoriale. Secondo, abbisogna di prestare attenzione alla ristrutturazione del sistema produttivo in costanza di fenomeni di macroeconomia e di natura e di natura sovranazionale che fanno sì che alcuni settori, che pure davano la possibilità di lavorare in questo come nei Paesi ad economia avanzata, oggi ahimè non ne danno più. Abbisogna di un ammodernamento e di una efficientizzazione della pubblica amministrazione, abbisogna di infrastrutture e di attenzione al sistema dei trasporti, perché ancora oggi aree del Paese come la Calabria, come la Puglia, vengono tagliate fuori, così come ahinoi accadde agli albori dello Stato italiano. La ricerca delle fonti energetiche, di fonti energetiche vere, che consentono di eliminare il *gap* del 30 per cento che noi abbiamo rispetto agli altri Paesi del maggior costo dell'energia. Ebbene, non si può dire che l'utilizzo del cosiddetto tesoretto, avviato per rivoli e rivoletti, come quello della riduzione dell'ICI, per alcune categorie e non anche per l'intera categoria della prima casa la sperata riduzione dell'aliquota IRES, per altro mimetizzata e vanificata da una diversa considerazione delle poste di interessi attivi e di ammortamenti anticipati che ne vanificano l'aspettativa, il credito per l'assunzione nel Mezzogiorno, ma chi vuoi che assuma nel Mezzogiorno, nelle aree deboli del Paese, laddove manca la sicurezza e la certezza per l'impresa, per la famiglia e per la persona? E qui veniamo all'altra emergenza, quella della sicurezza del vivere civile, che certamente deve essere coniugato con l'accoglienza, ma che non può essere vanificato con il permissivismo e con la possibilità per chi viene da fuori di non rispettare questo Paese. l'attenzione alla maternità, all'infanzia, alla gioventù, alla terza età, mentre viene eliminato l'arbitrato, un istituto che solo consente di ausiliare l'autorità giudiziaria inadeguata e non diciamo in questo momento per quali motivi, ma non certamente per colpa di magistrati, ad affrontare il problema della giustizia civile. E allora,

che la spesa corrente è aumentata, che la spesa pubblica supera il 50 per cento del PIL, non diciamo della pressione fiscale, che certamente laddove riteniamo di poterla ridurre per la categoria del lavoro dipendente, compiamo un'opera di diseducazione e di divisione del popolo italiano che non ha eguali: non possiamo trattare il lavoro dipendente diversamente dal lavoro autonomo, perché se è necessaria

e perché così com'è stato detto non emerge un progetto strategico nell'interesse del popolo italiano, noi daremo voto sfavorevole a questa vostra proposta di legge.

1818*. Signor Presidente, colleghe e colleghi senatori, i rari e rarefatti riferimenti alla legge di formazione del bilancio, disegno di legge n. 1818, ascoltati nel dibattito che si è sviluppato in queste due giornate in Aula, sono la spia di come, nonostante il lavoro fatto, il bilancio non sia ancora considerato strumento sufficientemente duttile

Tra il suddetto auspicio e la concreta realizzazione delle condizioni per il superamento della legge finanziaria, vi è ancora molto lavoro da fare, come si evince, per altro, dalla documentazione prodotta dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato negli ultimi mesi. È sulla persistente rigidità del bilancio, in particolare per ciò che concerne le scelte allocative della spesa, che occorre intervenire, persistendo nella sfida della trasparenza che - come ho cercato di argomentare nella mia relazione di ieri - sta conseguendo le prime vittorie. In conclusione, non posso che rinnovare l'invito a tutto il Senato della Repubblica ad offrire il proprio proficuo contributo affinché, sin dal prossimo gennaio, prosegua un serrato confronto istituzionale, finalizzato al trasparenza e dell'efficacia del bilancio di previsione dello Stato. tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione intervenuti: il dibattito è stato ricco e interessante. Naturalmente non vi è il tempo di replicare alle osservazioni formulate da molti, in particolare su temi specifici. Mi limiterò, in pochissimi minuti, a qualche battuta di replica sulle critiche di carattere generale, sull'impostazione della manovra finanziaria.

operato dalla Commissione, per di più senza copertura finanziaria. Queste affermazioni, che abbiamo ascoltato in questi giorni, in queste ore, sono generiche, talvolta pretestuose e, soprattutto, non supportate da alcuna specifica indicazione sulle presunte scoperture che si sarebbero verificate a seguito dell'approvazione di taluni emendamenti.

un aumento di spesa? Il senatore Vegas e gli altri intendevano dire che l'abolizione del *ticket* costituisce un aumento di spesa? Certamente no: non lo si può sostenere, tanto più che quell'intervento, com'è stato detto, trova ampia, puntuale copertura ‑ da nessuno confutata nel merito merito né contestata relativamente alle singole appostazioni di copertura ‑ attraverso appunto i tagli di spesa. Ma faccio anche altri due esempi, rapidamente.

O quelle risorse erano già destinate allo sviluppo del Mezzogiorno e sono state finalizzate su una misura che riteniamo di particolare efficacia? Oppure il pacchetto sui precari.

viene aumentato di soli 20 milioni di euro l'anno. Si opera un ampliamento molto contenuto sui requisiti soggettivi, sotto il profilo temporale della maturazione del diritto alla stabilizzazione; si conferma - e, se vi è bisogno di ulteriore precisazione, si può operare - la necessità delle procedure selettive. Quindi, anche in questo caso, dov'è dov'è la corsa alla spesa, la sanatoria generalizzata? Su un altro punto, Presidente, vorrei fare qualche battuta di replica. Si continuano a sostenere tesi come se, sotto il profilo della politica delle entrate, questa finanziaria costituisse il secondo tempo o la prosecuzione della finanziaria dello scorso anno: anche in È stato detto e lo sottolineo: questa è una finanziaria che non contiene nessun euro in più di nuove entrate; anzi, si orienta la pressione fiscale verso la discesa. Lo si fa con interventi organici di riforma per le imprese, per tutte, comprese le piccole; lo si fa anche per le famiglie con gli interventi specifici ricordati e che riguardano, per esempio, il settore della casa ed altri settori. Vogliamo o non vogliamo acquisire consapevolezza che stiamo operando verso la riduzione della pressione fiscale? Questa Questa è la domanda che vorrei porre ai colleghi. Infine, il tema anch'esso molto ricorrente negli interventi, che riguarda i risparmi, in particolare quelle riferiti ai costi della politica. In questi giorni, in queste ore, in quest'Aula e anche fuori, per la verità, c'è chi sostiene che abbiamo fatto troppo poco e c'è chi sostiene che abbiamo fatto troppo. Io credo che la verità stia nel mezzo, come spesso avviene: abbiamo fatto ciò che si poteva fare. Si può fare di più. Se il Governo stimerà, nei prossimi giorni, il complesso delle misure che sono state approvate, alcune molto innovative, si dimostrerà che il Senato ha operato interventi molto più incisivi di quelli originariamente prospettati e che si verificherà un risparmio sulla spesa pubblica molto consistente, da taluni ritenuto eccessivamente consistente. È la prima volta, signor Presidente, che il Parlamento, nel caso il Senato, fa sotto il profilo dei risparmi, del rigore più di quanto il Governo aveva proposto di fare. Ho concluso, Presidente. Devo dire la verità: nel dibattito, ma anche esaminando le proposte emendative, non ho ascoltato molte molte proposte alternative concretamente praticabili rispetto a quelle recate nella legge finanziaria al nostro esame.

non commendevoli, che dimostrano la non sostenibilità di una proposta alternativa rispetto a quella che abbiamo fatto, rispetto a quella che abbiamo esaminato approfonditamente in Commissione. Certamente ci sono ulteriori miglioramenti che quest'Aula e poi la Camera potrà apportare a questo testo, ma resto convinto del fatto che questa è una buona finanziaria, la migliore che si potesse fare in questo momento storico, sulla base di queste risorse e delle condizioni che ci sono date.

ho seguito il dibattito dagli schermi televisivi durante la mia giornata di lavoro al Ministero. La mia replica consisterà di breve considerazioni generali e di risposte specifiche ad alcune delle questioni sollevate. I disegni di legge finanziaria e di bilancio per il triennio 2008-2010 approdano all'Aula del Senato dopo una costruttiva discussione della competente Commissione. Rispetto allo scorso anno, è migliorata la struttura del disegno di legge finanziaria, che si presenta più snella nella forma e più ordinata nei contenuti. Specularmente al bilancio dello Stato, la finanziaria è ora strutturata per missioni, permette un'immediata valutazione delle risorse complessivamente disponibili per perseguire le finalità di pubblico interesse. La struttura non è certo perfetta, andrà forse modificata in alcune parti, ma, come ha sottolineato efficacemente la senatrice Menapace e come hanno sottolineato altri parlamentari, anche dell'opposizione, il Parlamento e il Governo sono ora in condizione di governare meglio gli eventi contenuti nei documenti finanziari. La Commissione bilancio ha lavorato, nelle scorse settimane, sul testo uscito dal Consiglio dei ministri. Sono stati rispettati i tempi, e di questo ringrazio il Presidente della Commissione e il relatore. Si è svolta una discussione pacata nei toni e costruttiva nei contenuti, che ha portato ad individuare alcuni qualificati emendamenti. Questi permettono di meglio soddisfare esigenze su cui il Governo, nella struttura originaria del disegno di legge, non aveva mostrato la stessa sensibilità della Commissione. Il passaggio parlamentare della manovra di bilancio è momento essenziale e non sostituibile della vita di una democrazia; procedure diverse, che pure sono presenti nelle esperienze di alcuni Paesi europei, non mi paiono da imitare. La manovra di bilancio viene preparata sempre, purtroppo, in maniera concitata. La mancanza della necessaria riservatezza e l'esiguità dei tempi impongono che il documento venga approntato prima che siano del tutto esaurite le necessarie interlocuzioni politiche e sociali. Il passaggio parlamentare permette allora una riflessione adeguata ed un dibattito approfondito, che favoriscono il miglioramento del documento. I problemi ai quali il bilancio e la finanziaria devono dare risposte sono molti, eterogenei, complessi; la maggior parte di essi ruota intorno al tema della crescita economica. Ho insistito più volte sulla sottocapitalizzazione del Paese, sulla necessità di interventi di politica economica che favoriscano gli investimenti produttivi e permettano una crescita economica più sostenuta. Ma non c'è crescita senza stabilità macroeconomica, senza conti pubblici sani e sostenibili. L'avanzo primario che si era azzerato nel 2005 si è riformato, raggiungendo nel 2007 il 2,5 Il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo ha ripreso a scendere e l'obiettivo di portarlo sotto il 100 per cento è a portata di mano: è questo il migliore investimento per il futuro. Un debito in calo significa minore spesa annua per interessi, più investimenti produttivi, la possibilità di ridurre la pressione fiscale sui cittadini che pagano onestamente le tasse. Il Paese ha poi bisogno di colmare un *deficit* di equità, che ha portato negli ultimi anni l'aumento della povertà relativa, che ha allargato il divario tra lavoratori stabili e precari, senza un adeguato sistema di tutele, che ha lasciato pressoché invariato il divario territoriale. Crescita, risanamento, equità: l'azione del Governo si muove lungo queste tre linee contemporaneamente e ciò rende complesso ogni disegno di legge finanziaria. Come ebbi modo di dire qui il 3 ottobre, è questo il modo per operare oggi guardando al futuro. Ma intervenire in maniera strutturale richiede tempo; non è una sola manovra finanziaria a poter risolvere difficoltà che si sono accumulate nel corso di anni. Sono direttamente impegnato nel migliorare la qualità della spesa pubblica. Circa 500 miliardi di euro sono iscritti nel bilancio pubblico sulla base delle leggi esistenti. La finanziaria rappresenta non più del 2-3 per cento di questa ingente massa di risorse. La finanziaria non è il solo strumento che può significativamente incidere. Servono una migliore programmazione delle risorse esistenti, una gestione orientata ai risultati, un'analisi e revisione critica dei programmi di spesa per riorientare le risorse - questo sì con la finanziaria - verso iniziative ritenute prioritarie. Vengo ora ad alcune osservazioni su punti specifici sollevati da onorevoli senatori durante il dibattito in Aula. Il senatore Maninetti osserva che il «Libro verde sulla spesa pubblica», da me presentato all'inizio di settembre, è rimasto lettera morta. Il Libro verde indica un percorso di innovazione culturale e amministrativa e un approccio diverso alla spesa pubblica: mostra che spendere meglio è possibile. Non mi meraviglio allora che in un mese il Libro verde non abbia dato pienamente i suoi frutti; mi meraviglio, invece, che nei cinque anni della legislatura precedente non si sia sentita la necessità di lavorare lungo la direzione del miglioramento della qualità della spesa. Il senatore Sterpa si augura di tornare alla legge di bilancio e di mandare in soffitta la finanziaria. Egli sa che questo è anche l'auspicio da me espresso durante l'intervento del 3 ottobre, ma il senatore Sterpa sa anche che questo è un cammino lungo. Il libro verde - spero che egli me ne dia atto - fornisce materiali conoscitivi indispensabili per muoversi in quella direzione. La manovra di bilancio esce dal lavoro svolto in Commissione intatta nella sua struttura e nei suoi interventi principali. Si confermano gli obiettivi per il 2008:

e ci fa sperare nella chiusura della procedura di *deficit* eccessivo. Ho notato con soddisfazione che diversi interventi in quest'Aula, tra i quali quelli del senatore Banti e del senatore Ria, hanno evidenziato l'importanza della ricostituzione dell'avanzo primario. primario. Al senatore Curto, il quale afferma - cito testualmente - che abbiamo "dilapidato i vari tesoretti determinati dalla politica virtuosa del precedente Governo", mi permetto di far osservare che quella politica non è stata virtuosa e che non vi è stata nessuna dispersione di risorse finanziarie nel 2007. Il decreto di luglio e quello di settembre hanno permesso di rimettere in moto le amministrazioni pubbliche, di anticipare spese per infrastrutture che andavano in ogni caso sostenute, di aumentare le pensioni minime e di onorare gli impegni in tema di aiuto allo sviluppo. Il senatore Martone ci ricorda gli alti impegni in tema di cooperazione allo sviluppo. Credo che gli interventi della finanziaria e del decreto-legge n. 159 che l'ha preceduta diano risposte importanti. In nessuno degli anni passati è stato fatto tanto quanto realizzato proprio in questi mesi. Il lavoro svolto sul testo del disegno di legge finanziaria nella Commissione bilancio, attraverso gli emendamenti approvati, ha rafforzato alcune componenti dell'azione di Governo e corretto, dal punto di vista tecnico, alcuni difetti, sempre presenti quando si predispone un documento complesso come la finanziaria. Vi è da parte mia un apprezzamento non formale al Presidente, al relatore e ai membri della Commissione per questo importante risultato. Nuovi incentivi all'occupazione nel Mezzogiorno; potenziamento delle dotazioni di risorse umane in alcuni settori strategici, come la lotta all'evasione, la tutela dell'ambiente; il funzionamento della giustizia; conferma, anche per il 2008, dell'abolizione dei *ticket* sanitari; incremento del fondo per le non autosufficienze: sono queste le principali misure uscite dalla discussione della Commissione che vanno nella direzione tracciata dall'azione del Governo di coniugare l'efficienza e il rigore con l'equità sociale. Tutte le iniziative contenute nel disegno di legge hanno copertura finanziaria, così come previsto dalla Costituzione. Si tratta più precisamente delle questioni attinenti l'impatto sul saldo netto da finanziare, che riguarda il bilancio dello Stato, così come previsto dall'articolo 81 della Costituzione. Le voci che si sono sollevate in questi giorni in merito a presunte situazioni di non copertura - e mi riferisco in particolare all'emendamento che ha prorogato la sospensione fino a tutto il 2008 del *ticket* sull'assistenza ambulatoriale specialistica di 10 euro - sono favole strumentali e poco responsabili. Riguardano più propriamente la stima degli effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, che è un aggregato statistico. Ricordo all'Assemblea che l'effetto di qualsiasi provvedimento finanziario sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è materia di stima, non è un dato certo, in quanto lo stesso concetto di indebitamento netto è una costruzione statistica basata su convenzioni internazionali. Il *deficit* che si è creato nella scorsa legislatura e l'abnorme differenza tra fabbisogno di cassa e indebitamento netto che è stata evidenziata nella passata legislatura da parte di istituzioni nazionali ed internazionali sono la prova di quanto le stime possano essere fallaci. Abbiamo trovato un dissesto dei conti pubblici; stiamo faticosamente operando per correggerlo.

Dicevo che abbiamo trovato un dissesto dei conti pubblici e che stiamo faticosamente operando per correggerlo. Mi pare che il concetto sia chiaro. Ho letto alcune insinuazioni di stampa. Con la Ragioneria generale dello Stato, uno dei quattro Dipartimenti in cui si articola il Ministero dell'economia e delle finanze, c'è un'intensa e proficua interlocuzione,

e per questo ritengo superfluo ripercorrere tutto il disegno di legge. Cito solo alcuni punti sui quali la Commissione è intervenuta con miglioramenti. Inizia la restituzione fiscale: l'aumento della detrazione ICI sulla prima casa, il *bonus* per i soggetti a basso reddito e i loro familiari, le diverse agevolazioni fiscali predisposte con la manovra sono possibili grazie all'azione di contrasto all'evasione fiscale. Sono d'accordo con la senatrice Pellegatta che il potenziamento della lotta all'evasione è un'importante innovazione introdotta nel testo originario della finanziaria. Va poi ricordato l'importante emendamento approvato dalla Commissione, che destina l'eventuale gettito aggiuntivo alla riduzione della pressione fiscale sui lavori dipendenti. Il disegno di legge finanziaria fornisce anche una prima risposta, forse ancora parziale, alla riduzione dei costi della politica. Il lavoro in Commissione ha introdotto la riduzione del numero dei membri del Governo in modi e forme compatibili con la Costituzione ringrazio il senatore Villone per averlo ricordato in quest'Aula. Anche le modifiche apportate dalla Commissione ad alcune norme, in particolare quelle sulle comunità montane, hanno mantenuto il senso complessivo degli interventi, malgrado ciò che ha affermato questo pomeriggio il senatore Saia. Il tema dei costi della politica è complesso e differenziato - come ha sottolineato il senatore Perrin non tutti i costi sono sintomo di inefficienza: questo vale per i consigli circoscrizionali, per le indennità parlamentari, per il numero dei consiglieri comunali. Sottolineo, per inciso, che l'intervento proposto dal Governo e perfezionato dalla Commissione in merito alle Comunità montane ha l'obiettivo di ridurre i costi impropri delle strutture per destinare i risparmi in favore dei territori montani, attraverso l'aumento del Fondo per la montagna; fondo che era stato prosciugato nel corso della precedente legislatura. Per lo sviluppo del Mezzogiorno, utilizzando risorse già stanziate con il Fondo per le aree sottoutilizzate, l'emendamento approvato in Commissione prevede per il 2008 un credito d'imposta per l'assunzione a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, superiore ai 4.000 euro l'anno per lavoratore e queste somme diventano quasi 5.500 euro l'anno nel caso di assunzione di donne: rispettivamente, oltre 330 euro al mese e oltre 415 euro al mese. L'utilizzo di strumenti automatici riduce la burocrazia connessa all'erogazione discrezionale di incentivi, pone tutte le imprese sullo stesso piano, permette la crescita dell'occupazione a tempo indeterminato, soprattutto delle donne. Va anche ricordata l'aumentata efficienza dell'utilizzo delle risorse, facendo confluire quelle del FAS nel quadro strategico nazionale e attivando - lo sottolineo - 100 miliardi di euro fino al 2013. Vi è poi il capitolo sicurezza, tema che è al centro del dibattito nel Paese in questi giorni. La finanziaria interviene stanziando risorse aggiuntive per i Carabinieri, per la Polizia di Stato, ma anche per chi opera a tutela del territorio e dell'ambiente: i Vigili del fuoco e il Corpo forestale dello Stato. È chiaro che senza risorse finanziarie non si fa lotta alla criminalità e il Governo ha mostrato, nei limiti dei vincoli di bilancio, un impegno e uno sforzo straordinari; inoltre, la stessa Commissione bilancio ha rafforzato e incrementato le risorse disponibili. è altrettanto certo che la lotta alla criminalità richiede anche, come tutti i settori della pubblica amministrazione, un continuo sforzo per individuare le migliori pratiche che si realizzano quotidianamente nell'operare delle forze dell'ordine e applicarle a tutte le realtà diffuse diffuse nel territorio. Infine, vorrei sottolineare l'attenzione alle problematiche dell'ambiente. Una politica economica che guarda al futuro deve tutelare le proprie risorse naturali e ambientali. Tra le iniziative contenute nel disegno di legge finanziaria ricordo la conferma degli stanziamenti per Kyoto, la creazione di nuovi parchi urbani, le misure per il contrasto al dissesto idrogeologico, gli ampi sgravi fiscali per le spese di ristrutturazione delle abitazioni secondo criteri di ecoefficienza. In quest'ambito rientrano anche gli interventi citati dalla senatrice Donati per migliorare la mobilità dei centri urbani. Sono risposte concrete a esigenza non più procrastinabili di una migliore qualità dell'ambiente. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo ha attentamente ascoltato i lavori di quest'Aula e ne ha apprezzato i toni costruttivi da parte sia delle forze di maggioranza sia di quelle di opposizione. Credo che questo sia segno di piena consapevolezza del Parlamento, del cambiamento in corso nel Paese, della fine della contrapposizione ideologica e della forte richiesta che viene dai cittadini di dare risposte concrete e tempestive a problemi reali. I disegni di legge finanziaria e di bilancio in discussione sono tasselli dell'azione intrapresa dal Governo per il risanamento economico, per ridurre la disuguaglianza sociale, per garantire una crescita del Paese sostenibile oggi e nei prossimi anni. Abbiamo coniugato le molteplici esigenze del Paese guardando all'oggi, ma non meno al domani. Non abbiamo moltiplicato i pani e i pesci. pesci. Più modestamente abbiamo cercato di usare nella maniera più ragionevole le risorse disponibili. Spero che il Parlamento lavori per migliorare ulteriormente il testo uscito dalla Commissione bilancio, nel rispetto dei tempi previsti

*(AN)*. Signor Presidente, come avvenuto nel dicembre del 2006 per il 2007, quando il Governo nascose 26 miliardi di entrate facendole emergere nel corso di quest'anno solo parzialmente e chiamandole tesoretto, per poi disperderle in flussi di spesa pubblica (ma è tutto quello che ci siamo detti in quest'anno), ebbene, c'è una reiterazione di reato anche per il 2008. quindi che nel bilancio dello Stato per il 2008 venga appostata la cifra giusta, sulla base dei dati ufficiali del Governo. Dati ufficiali che devono partire dal preconsuntivo 2007, moltiplicato per la crescita economica prevista dal Governo e per l'elasticità entrate-PIL dichiarata dal Governo. Con queste due semplici moltiplicazioni si ottiene una cifra di entrata che è almeno 14 miliardi superiore a quella che il Governo ha iscritto a bilancio. Delle due l'una, signor Presidente e onorevoli colleghi: o il Governo scrive le cifre giuste sul bilancio per il 2008 sulla base dei suoi stessi dati contabili oppure il Governo deve dichiarare che le previsioni di crescita fatte a settembre oggi sono sbagliate, che la crescita è inferiore e che quindi le entrate potrebbero essere inferiori. Ma se la crescita rimane la stessa, mancano ad iscrizione a bilancio 14 miliardi.

da esse egli deriva previsioni finanziarie che si discostano da quelle del Governo e della maggioranza.

e che è stato l'obiettivo di finanza pubblica perseguito da tutti i Governi europei negli ultimi quindici anni, non è un dato di finanza pubblica ma un semplice aggregato statistico.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Ministro, la sua replica non ci ha convinto. Finalmente abbiamo potuto ascoltarla direttamente, dopo le sue estemporanee esternazioni dei giorni scorsi, non nelle sedi parlamentari ma in occasione di contatti con i media che lei privilegia. Ma non è su questo che voglio parlare. Voglio soffermarmi sulla sua recente affermazione che le tasse sono bellissime:

Che le tasse siano bellissime forse è dovuto al suo eccezionale senso estetico; il problema a questo punto non è se sono bellissime, ma l'uso che di esse si fa e voi ne state facendo un uso così apprezzato dai nostri cittadini contribuenti che sono finiti in massa a sostenere le sparate di Beppe Grillo, che hanno alimentato l'antipolitica e la cultura delle caste.

non sono solo quelle degli uomini delle istituzioni ma anche del mondo dei media. A questo punto dobbiamo ringraziare l'ottimo lavoro del Servizio studi del Senato, che ha illuminato di immenso, come avrebbe detto Ungaretti. Tremonti ha provocatoriamente detto, non senza fondamento, che l'esercizio provvisorio sarebbe positivo per i conti pubblici, tant'è che i saldi programmatici sono peggiori del dato tendenziale, che quella sarebbe la migliore finanziaria. Condivido, allora, quanto affermato ieri da Nicola Rossi sulle colonne di un grande quotidiano nazionale, di risparmiarci le prediche, perché lei non ha mancato di farci un'ulteriore predica. È questa l'utilità di spendere i tesoretti - ammesso che esistano sul serio - di fronte ad un debito pubblico in crescita in valori assoluti come quello italiano? In tutto il mondo, quando si è voluto combattere l'evasione e portarla a livelli fisiologici si sono abbassate le aliquote,

si è provveduto contestualmente a ridurre le spese correnti e quindi si è ridotto il fabbisogno mensile e lo *stock* di debito. Tutto il contrario - non rida, signor Ministro - di quanto avete fatto voi che avete dilapidato queste maggiori entrate fiscali. una lettura attenta delle entrate non porta alle conclusioni della sua relazione, un misto di filosofia mal digerita. Le conclusioni sono ben altre, infatti, perché non ha tenuto conto di questi elementi. La relazione contiene una stima del sommerso del 18 per cento che appare ottimistica. Se la Banca mondiale stima in 300 miliardi l'anno il sommerso italiano, ne deriva che sarebbe ben superiore. I 23 miliardi di maggiori entrate da recupero dell'evasione introitati nel 2006-2007 appaiono pertanto una percentuale ancora troppo esigua rispetto all'ammontare complessivo. Le entrate tributarie della pubblica amministrazione sono cresciute del 3,1 per cento nel 2005 e del 10 per cento nel 2006. Occorre però leggere in modo corretto tale incremento. Infatti, analizzando l'andamento recente della crescita economica, si nota, nel 2005, la presenza di un dato anomalo, con un tasso di crescita del PIL molto basso, pari allo 0,2 per cento, mentre riportandosi sui valori in linea degli anni precedenti al 2005. Ne consegue, signor Ministro, che la variazione 2006 sul 2005 delle poste fiscali risente in misura notevole di questo forte recupero della crescita 2006 rispetto alla fase di stanca dell'anno precedente. Il 2005 rappresenta la peggiore *performance* di crescita degli anni 2000. Usarla quindi come base di calcolo diventa fuorviante. Il recupero del PIL nel corso del 2006 contiene una ripresa sufficientemente sostenuta dei consumi delle famiglie, il che può avere innescato una pressione sulla domanda aggregata. Come conferma di questi andamenti, nel 2006 l'inflazione misurata dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo è stata superiore al deflattore implicito del PIL (2,2 contro 1,8). Pertanto, il carattere di eccezionalità dell'aumento delle entrate tributarie è in parte dovuto ad un rigonfiamento dei valori nominali. Il positivo andamento delle entrate tributarie ha caratterizzato anche gli altri Paesi europei

Se osserviamo tuttavia i dati relativi alla crescita economica nel 2005 e nel 2006 negli stessi Paesi, rileviamo che in Germania si è passati dallo 0,9 al 2,7 per cento, in Francia dall'1,7 al 2 per cento, in Spagna dal 3,5 al 3,8. L'entità degli incrementi delle entrate sembra dipendere fortemente dalla dinamica del ciclo economico, dato che le maggiori variazioni sulle entrate si sono registrate nei Paesi che hanno avuto un forte incremento di crescita, come la Germania. Se, inoltre, teniamo conto della maggiore inflazione italiana rispetto alla Francia e alla Germania, quantificabile in 30-40 punti base, il dato di una migliore *performance* italiana nel confronto europeo non appare così evidente. Il gonfiamento delle basi imponibili dovuto all'inflazione non è mai menzionato nel suo documento, quando invece ha un ruolo importante nel determinare il gettito. La restituzione del *fiscal drug* riporterebbe il gettito su livelli fisiologici per le famiglie italiane e ridurrebbe l'azione redistributiva tra i contribuenti onesti e quelli opportunisti. Inoltre, va ricordato come il gettito proveniente dalla lotta all'evasione sia puramente contabile: gli incassi provenienti dai ruoli, cioè l'effettivo introito di cassa, derivante dal processo di accertamento fiscale, misurano solo un residuo contabile tra bilancio di competenza e di cassa. Ad oggi, l'Agenzia delle entrate non è in grado di stabilire l'effettiva entrata di cassa proveniente dagli accertamenti fiscali. Occorre allora un migliore coordinamento all'interno dell'Agenzia e tra Agenzia e Ministero, per stimare gli effettivi introiti derivanti dalla lotta all'evasione, i tempi di riscossione e la percentuale di crediti in sofferenza. In conclusione, signor Ministro, la *performance* italiana sul gettito tributario 2006 è sovrastimata, in seguito ad un effetto nominale che incide maggiormente sulle entrate tributarie rispetto al PIL, ad un gradino di crescita nel passaggio dal 2005 al 2006, che incide sulla dinamica delle entrate in misura preponderante rispetto ad un effettivo recupero dell'evasione e - nel confronto internazionale - ad una maggiore inflazione italiana, di cui lei non ha tenuto conto. Per queste ragioni e considerazioni, esprimo il netto voto contrario sulla Tabella dell'entrata, perché mi rifiuto di prendere in giro gli italiani attraverso frasi ad effetto e demagogiche come quella da lei pronunciata, quando ha sostenuto che le tasse sono bellissime.

dei criteri che ci hanno guidato alla compilazione di questi emendamenti. Volevamo verificare per via emendativa se effettivamente fosse vero che la cosiddetta nuova struttura del bilancio avrebbe portato una migliore conoscenza e anche un migliore grado di emendabilità, in sede parlamentare, delle relative appostazioni. Il lavoro che abbiamo svolto consiste nella

per le singole missioni. Ma in realtà, facendo questo lavoro, abbiamo scoperto che un po' pirandellianamente tutto è cambiato perché nulla cambiasse. Infatti, se guardiamo alla sostanza, sono rimaste vecchie unità previsionali di base, ancorché distribuite in modo diverso, ma il limite di emendabilità contenuto nel bilancio è stretto esattamente come prima.

sarebbe indispensabile per realizzare veramente una differenziazione per funzioni o per missioni della spesa pubblica, per consentire al Parlamento e ai cittadini di capire se è più importante sviluppare, ad esempio, la spesa nel settore della difesa rispetto a quella dell'istruzione o viceversa. Ciò non è consentito con questo tipo di bilancio. Questo è il il frutto dell'esercizio che abbiamo compiuto, che dimostra come ancora una volta la parte manovrabile è modestissima, la finanziaria lavora al margine per entità risibili rispetto al complesso della spesa pubblica e quindi tutto l'insieme del meccanismo è poco

l'amministrazione pubblica nel suo complesso. Se non si interviene con strumenti nuovi e diversi, non riusciremo a risolvere i più importanti problemi di funzionamento dello Stato. Detto questo,

negli ultimi mesi con la cosiddetta *spending review*, operazione credo più di immagine che di sostanza. Infatti, quando si fa un'analisi di carattere finanziario-economico delle spese di bilancio certo si aggiungono elementi conoscitivi, ma manca l'elemento fondamentale, un elemento di carattere giuridico, perché il nostro bilancio lavora sulla base di autorizzazioni legislative, che costituiscono quasi il 90 per cento del complesso della spesa. La *spending review,* per avere un senso, deve essere impostata sulla ricognizione degli effetti quantitativi e finanziari delle disposizioni legislative e, sulla base di queste, intervenire per modificarle o per cancellarle. Bisogna quindi arrivare a una sorta di clausola di *sunset legislation*, di legislazione del tramonto, nella quale si delinea anche la fine dell'efficacia di norme giuridiche,

dall'appartenenza alla maggioranza o all'opposizione. Infatti, come si è dimostrato, dopo tutte le finanziarie ci si lamenta dell'incapacità dello strumento di essere utile al Paese ed ogni anno si ripetono gli stessi errori.

Come ricordava il senatore Vegas, siamo di fronte a un esercizio teorico del quale non sottovalutiamo l'interesse né i risultati empirici. Nella proposta non ci è sfuggita nemmeno la rilevanza politica di alcuni emendamenti. Vorrei ricordare all'Assemblea che la Commissione, in effetti, ha accolto alcuni emendamenti presentati al bilancio, dei quali vorrei segnalarne almeno uno per importanza. Il più significativo riguarda lo spostamento di 10 milioni di euro dal programma dei servizi istituzionali e generali del Ministero dell'economia e delle finanze a quello del Ministero dell'interno, per ciò che concerne la missione ordine pubblico e sicurezza. Voglio anche sottolineare come la Commissione abbia condiviso una scelta fuori da ogni logica emergenziale. In maniera simile, altri tre emendamenti dell'opposizione, che sono più un segnale politico che la Commissione ha voluto dare al Governo e a tutto il Senato, essendo molto scarsa la loro rilevanza economica, hanno riguardato un appostamento di cifre maggiori sui capitoli che riguardano la tutela della salute, della ricerca scientifica di base e della ricerca universitaria. Questa breve premessa mi è servita per

Interverremo soltanto su quelle che sono le nostre proposte più significative, ma è chiaro che per quanto attiene al contrasto al crimine, nei giorni

per quanto riguarda questo stanziamento, che chiediamo di aumentare, vorrei porre all'attenzione sia del relatore sia del Governo la nostra necessità di incrementare i nostri fondi a favore della regolamentazione e della vigilanza del settore finanziario. Non voglio dilungarmi sul tema della finanza derivata, che ci sta tormentando in questi giorni, in quanto pone alla nostra attenzione la gravità

del relatore e del Governo non tengano assolutamente conto della nostra proposta e nell'articolato della finanziaria non ci sia nulla che faccia riferimento a questo importante problema, che è stato sollevato recentemente nel nostro

funzione primaria del Dicastero, che è quella del servizio universale e, quindi, della consegna della corrispondenza: a causa di questa deriva ci sarebbe una profonda alterazione della concorrenza. Che significa, infatti, questa appostazione? Desidererei una risposta da parte dell'Esecutivo nel merito di una decisione che apposta risorse per una liberalizzazione che non produce risparmi, bensì maggiori costi per la collettività.

Governo rispetto al quesito che avevo posto; altrimenti, facciamo una maratona senza significato. C'è un dovere del Governo di rispondere agli interrogativi posti.

Signor Presidente, gli emendamenti 22.1 e 22.2 sono diversi dagli altri. Essi mirano a sopprimere due commi nei quali vi sono conservazioni di residui. So che è una pratica utilizzata anche in passato, tuttavia, la conservazione dei residui va contro il principio dell'annualità del bilancio. Sarebbe meglio in questa azione di pulizia abbandonare anche le vecchie prassi e cercare di stanziare in bilancio quello che effettivamente è spendibile nel corso dell'anno, senza consentire pratiche che

ha detto che l'emendamento sui *ticket* è coperto; noi, invece, assistiamo ad una scopertura, perché non c'è la bollinatura della Ragioneria. È bene che la Presidenza e il Governo chiariscano questo aspetto prima della seduta di domani.